nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Sull'ordine dei

il parere della Commissione bilancio, di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul subemendamento 1.0.500/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.118, 1.119, 1.0.113, 1.0.114 e 1.0.115. 1.0.115. Il parere è di nulla osta sulle proposte 1.0.500, 1.0.500/2 e 1.0.500/3».

delle semplificazioni rispetto alle piccole difformità esistenti negli edifici colpiti dai danni del terremoto e che in questo momento bloccano buona parte delle ricostruzioni. Ci riferiamo a interventi fino alla manutenzione straordinaria con rilevanza strutturale: vengono quindi accorpati accorpati i procedimenti alla domanda di contributo, c'è una semplificazione rispetto alla normativa per quanto riguarda l'autorizzazione sismica e, ovviamente, in caso di vincolo paesaggistico, c'è l'assoggettabilità alla alla conformità ambientale, con procedimento semplificato. Si tratta di un primo passo verso la soluzione di un problema che è stato segnalato da tanti sindaci, da tanti amministratori locali e dai cittadini. In cercare quella soluzione azzeccata di cui parlava il Presidente della Regione Abruzzo nelle sedute precedenti.

Non concordiamo neppure sul fatto che non ci sia la copertura finanziaria, perché evidentemente il problema è risolvibile nel momento in cui si modificano i criteri. Insistiamo quindi per la votazione dell'emendamento.

sollecitato e concerne una problematica di cui ci si è accorti in maniera massiccia in corso d'opera e recentemente, nelle ultime settimane. alle piccole difformità di tipo edilizio e urbanistico che sono molto diffuse, spesso non eliminate per la mancanza di piani urbanistici comunali, e che

con intenti speculativi o ipotesi ancora peggiori. Si tratta, quindi, di piccole difformità su cui tutti quanti abbiamo detto che è necessario intervenire. Voglio anche dire che c'è stato un lavoro preparatorio che la commissaria straordinaria

giungere a un risultato più forte e ampio, ma condiviso da tutti, su questo tema, che è decisivo, altrimenti l'*iter* della ricostruzione non si completerà

la parte di aziende che hanno avuto oggettivamente un danno. Tale è l'impegno che oggi voglio comunicare a questo ramo del Parlamento.

intervengo sulle dichiarazioni del Governo.

La ringrazio, signor Presidente; lei mi consentirà di non essere d'accordo con la sua interpretazione, ma la ringrazio comunque, perché è lei che decide in questo caso. A me pare francamente che le dichiarazioni

Detto in altri termini, i soldi arrivano dove ci sono condizioni perché questi possano fruttare. Il Governo si dovrebbe rendere conto

terribili. Come si fa a considerare quelli come aiuti di Stato non leciti? Il Governo dovrebbe dire con chiarezza che quegli

la restituzione di questi soldi provocherà l'uscita dal mercato di una serie di aziende che miracolosamente erano riuscite a rimanervi dentro, se provocherà disoccupazione, questo sarà un modo per applicare ciò che avete detto ieri o sarà un modo per contraddirlo? Infine - l'ultimo e più importante punto non ha mai detto e scritto che la decisione sul *de minimis* è aiuto di Stato. Nella lettera inviata al sindaco Biondi si dice una cosa diversa, quindi il parere

poiché siamo persone ragionevoli e riteniamo che gli interessi dell'Aquila siano più importanti di qualsiasi speculazione politica, noi siamo disponibili ad accedere a qualsiasi soluzione. Ma a condizione che vi sia un impegno chiaro: che il problema venga risolto entro il tempo di questo decreto-legge. I due mesi da soli non bastano, anche perché uno sarà il mese di agosto e quindi servirà semplicemente a rendere la ferita più purulenta. *(Applausi dal

di grande rilevanza, come diceva il collega Quagliariello, perché riguarda moltissime imprese dell'Aquila. Se non interveniamo - dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile; dobbiamo farlo

Noi dobbiamo assolutamente intervenire. La proroga approvata in Commissione speciale l'abbiamo votata, ma con l'auspicio che in Aula potessimo fare di più. Per questo manteniamo questo emendamento. Tra l'altro, la commissaria europea competente si è già espressa chiaramente nel merito di questa materia,

rispetto al quale il Governo ha fornito dei pareri, dei chiarimenti e alcuni approfondimenti. Come ha fatto il collega Quagliariello, intendo motivare la nostra posizione rispetto a questo emendamento. Abbiamo anche dato la disponibilità - lo ha anticipato prima il senatore Quagliariello - a individuare di comune accordo una possibile transizione. Naturalmente, se c'è l'intenzione di porre in votazione l'emendamento noi, e sul merito, voteremo a favore del nostro emendamento e, quindi, a quel punto resta in discussione.

dal Ministero per ottenere documentazioni e carte che parlino in maniera più chiara delle eventuali ragioni sia stato poco fruttuoso. È una responsabilità che non riguarda solo il Governo in carica da qualche giorno, anche il Governo in carica precedentemente non è stato in grado di rispondere a un'iniziativa sbagliata e ostile dell'Europa e rispetto alla quale, negli uffici dei Ministeri competenti, c'è stata troppa arrendevolezza. Anche nella risposta portata in Commissione bilancio si affermano in maniera apodittica delle valutazioni. Ad esempio, si dice che si è in presenza di un dato testuale contrario e di un espresso diniego della Commissione europea al fatto che il *de minimis* sarebbe applicabile nel quadro temporale del 2011, cioè a 500.000 euro, e che anche l'emendamento subordinato, la norma d'interpretazione autentica, che potremmo adottare e che abbiamo presentato come subordinato all'emendamento del *de minimis*, sarebbe stato negato in presenza di questo dato testuale. Noi però non abbiamo nessun dato testuale. rappresentato alle amministrazioni locali, cioè al sindaco dell'Aquila e al governo della Regione Abruzzo, è sempre stato riferito in maniera verbale. Invito il Sottosegretario da questo punto di vista a fare un ulteriore approfondimento nei giorni che seguiranno. Inevitabilmente la questione si andrà trascinando, e a far tirar fuori dal Ministero anche questi presunti e autodichiarati dati testuali, secondo i quali l'Europa avrebbe già già risposto negativamente all'Italia sul fatto che il quadro di riferimento temporale da applicare è quello dell'entrata in vigore della norma e non della sua decorrenza

Cerco di spiegarmi. Qui in Aula il Governo si deve assumere un impegno definitivo, entro luglio, a risolvere questo problema e la strada principe è quella che diceva il collega che mi ha preceduto, vale a dire riportare la soglia dei 500.000 euro, che è il *de minimis*, stabilito allora, dell'Unione europea e non deciso da noi. Questo risolverebbe il problema, tant'è che avevo anche ipotizzato una correzione dell'emendamento proprio per dire questo. In ogni caso, se ci fosse un impegno dell'Esecutivo e tutta l'Assemblea fosse convinta, di fronte a questo impegno del Governo, a non andare al voto, allora staremmo tutti sull'impegno del Governo. Diversamente, se si dovesse andare al voto, noi voteremo questi emendamenti.

Se da parte del Governo c'è un impegno preciso, così come evidentemente lei auspica, io credo che ci sarebbe la disponibilità di tutta quanta l'Assemblea.

al Governo italiano, il problema è risolto. È semplicemente un problema interpretativo, che non implica nemmeno considerazioni di bilancio, perché saremmo tutti d'accordo - e anche l'Europa dovrebbe prenderne atto - che se l'interpretazione è quella secondo la quale la misura rientra nel termine del 2011,

analogo a quello presentato in quella sede e che - lo sottolineo - è stato approvato all'unanimità. Qualcuno mi potrà obiettare che ripresentare un analogo ordine del giorno può essere superfluo; in realtà, quest'ordine del giorno chiede sostanzialmente due cose al Governo: impegnarsi intraprendere con le istituzioni europee, in particolare con la Commissione, una negoziazione in ordine alla procedura d'infrazione che è stata avviata; e, e, nelle more di queste interlocuzioni, valutare l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni, ad oggi fissato al 22 luglio,

l'Assemblea ieri ha approvato un emendamento del relatore Patuanelli, l'1.0.2.000, che chiedeva - e ha ottenuto - la proroga di due mesi della presentazione delle osservazioni. Tenuto conto che la conversione del decreto potrebbe arrivare a ridosso della data del 22 luglio, magari uno o due giorni prima o due o tre giorni dopo, ritengo opportuno che il Governo, qualora dovesse emanare

di esprimere parere favorevole e quello che rivolgo a tutta l'Assemblea è di sostenere all'unanimità questo ordine del giorno, che diventerebbe un ulteriore vincolo per il Governo rispetto agli impegni testé illustrati dal sottosegretario Castelli.

A questo punto, prima di procedere al voto dell'ordine del giorno, chiedo al senatore Verducci e al senatore Marsilio se vogliono sottoscriverlo e ritirare i propri emendamenti oppure se intendono mantenerli.

UV))*. Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore del provvedimento e auspica una rapida approvazione da parte della Camera. È un atto doveroso nei confronti delle 600.000 persone che abitano nelle zone colpite dal terremoto e di un territorio che, come ha ricordato il relatore, conta 138 Comuni, 340.000 abitazioni e un tessuto sociale e produttivo di grande importanza. Abbiamo apprezzato il lavoro che tutti i Gruppi hanno condotto in Commissione speciale. È fondamentale che su temi come questo vi sia unità di intenti da parte di tutte le forze politiche. In questi casi non c'è colore politico che tenga; ci sono le istituzioni, in cui tutti lavorano con il massimo impegno. Sul merito delle questioni, signor Presidente, siamo d'accordo sulla necessità, espressa dal relatore, di dar vita a una guida interpretativa per superare le incertezze e i problemi creati dalla costante produzione normativa. La stratificazione delle norme rischia di tramutarsi in un ostacolo burocratico per la ricostruzione e per le misure a beneficio delle famiglie e delle imprese: un tema, questo, evidenziato anche dal commissario straordinario. Durante le audizioni in Commissione speciale, Confindustria ha portato un articolato per una legge quadro sulla gestione delle emergenze. È un tema importante, su cui sarà necessario intervenire per migliorare l'efficacia degli interventi e affrontare in maniera organica tutto quello che, nell'emergenza, poi si tramuta in un dilemma normativo. Pensiamo agli aspetti legati allo smaltimento delle macerie, alle proroghe fiscali, alle misure di sostegno per il tessuto produttivo: tutti aspetti che possono essere oggetto di una legge quadro, dalla quale determinare risorse e tipologie di misure, naturalmente a seconda della specificità delle situazioni e della loro gravità. In ogni caso, l'elemento più importante del decreto-legge è la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza. In questo modo, la prossima legge di bilancio potrà essere il sicuro terreno per lo stanziamento delle risorse ancora necessarie per la ricostruzione. In conclusione, colleghe e colleghi, crediamo che in nessun modo si debba abbassare l'attenzione per quelle zone d'Italia che hanno patito eventi

Presidente, colleghe e colleghi, come già molti hanno sottolineato nel corso della discussione generale, siamo di fronte alla più grande emergenza degli ultimi anni: nove scosse di magnitudo superiore a cinque, grande distruzione, dimensione territoriale inedita nella storia dei terremoti. questi terremoti si inseriscono all'interno di un territorio già profondamente compromesso - forse di questo bisognerebbe avere maggiore consapevolezza

non solo per i vincoli, ma per il dramma dell'assetto idrogeologico. Siamo di fronte a Comuni, nei quali il processo di spopolamento, prima del 24 agosto 2016,

hanno spesso segretari comunali "a scavalco" su due Comuni, se non su quattro. Molti Comuni hanno il sindaco, un vigile urbano e, quando va bene, il segretario a scavalco e un tecnico. Ho visto, nella mia esperienza, Comuni nei quali non si faceva una gara da circa otto anni per le condizioni strutturali di quei Comuni, con delle conseguenze: in otto anni le norme sulle gare sono cambiate radicalmente. Se poi andiamo a vedere la debolezza strutturale dei servizi, ci accorgiamo che in quelle aree una delle infrastrutture più moderne è forse la Salaria, che hanno costruito i romani. Tutto questo ha messo in condizioni veramente difficili il processo di gestione dell'emergenza prima e di ricostruzione Sarà bene avere questa consapevolezza, come abbiamo visto anche nel lavoro della Commissione. Io ringrazio qui il relatore e ringrazio tutti i Gruppi. Abbiamo fatto un lavoro secondo me positivo. di questo provvedimento. Avete visto che il nostro comportamento è stato coerente con gli impegni e con il lavoro svolto in Commissione; ma è bene avere questa consapevolezza. l'emendamento che abbiamo testé votato sulle piccole difformità o i piccoli abusi - non dobbiamo avere paura delle parole ci dimostra quanto ciò sia complicato. I colleghi della Commissione speciale sanno che avevamo trovato insieme una soluzione, che consideravamo positiva. Tuttavia, gli apparati dei Ministeri ci hanno detto di no. È un percorso noto è molto più semplice fare annunci o critiche; è più complesso il processo di costruzione reale delle norme. Lo dico non in senso polemico, come credo sia ben comprensibile, ma per spiegare qual è livello di difficoltà in cui ci si trova. Ho già detto che noi voteremo questo provvedimento convintamente e apprezzando il lavoro fatto, anche il lavoro del Governo, nonostante il Governo ci abbia detto no, assumendosi però degli impegni, che poi cercherò di riassumere, su una serie di questioni. Vorrei, però, approfittarne per cogliere una sollecitazione del relatore e alcune richieste che sono emerse anche da alcuni interventi, soprattutto dei colleghi senatori del MoVimento 5 Stelle. La prima è del relatore. Il relatore si è chiesto se è possibile costruire un provvedimento generale sul tema delle grandi emergenze e delle grandi catastrofi. Io sono pienamente d'accordo. Lo dovremmo fare; è indispensabile farlo. Consapevoli del fatto che ogni terremoto ha la sua dinamica: una cosa è un terremoto che avviene in pianura ed una cosa è il terremoto del Centro Italia, che avviene in un territorio difficile e già compromesso. Tuttavia, occorre affrontare alcune questioni. Così, voglio dirlo ai colleghi che hanno sollevato questo tema. Penso che dovremmo partire dall'analisi, senza strumentalizzazioni politiche, delle esperienze dei terremoti che ci stanno alle spalle: dal Friuli, alle Marche e all'Umbria, all'Aquila, all'Emilia e adesso al Centro Italia. Guardiamole queste esperienze, valutiamole perché, al di là di quanto ci diciamo negli interventi, le cose reali si vedono.

bisogna che definiamo che cos'è «emergenza» e che cos'è «ricostruzione». Definiamolo, onde evitare che, in modo pendolare,

non può esserci un meccanismo di interpretazione. Per capirci, visto che non voglio sfuggire al problema, quello che è successo a Norcia, già precedentemente ricordato, a proposito di una struttura temporanea, donata e finalizzata alla tutela a fronte del rischio di ulteriori terremoti, di tenuta strategica. Non può esistere un'interpretazione diversa, ma questo non può essere lasciato in mano - diciamo così - al buon spirito di questa o di quella componente dello Stato: deve trovare invece una risposta normativa.

Bisogna trovare una forma per costruire un coordinamento tra le normative finanziarie e di bilancio e la scelta politica degli interventi che lo Stato vuole compiere. Non si può infatti scrivere in una norma di bilancio «fino all'esaurimento dell'emergenza», perché è chiaro che il problema non sarà risolto. Dunque, c'è un grande e interessante lavoro da fare, ma senza la consapevolezza di una distinzione tra ricostruzione ed emergenza non andremo da alcuna parte.

di una scelta nuova, che non può essere riprodotta in tutti i territori, perché è chiaro che se fosse applicata in una grande città

È, quindi, determinante. In terzo luogo, c'è un credito d'imposta che assicura la ricostruzione. Non tutti gli anni i privati dovranno chiedere il rifinanziamento, perché il meccanismo è assicurato.

nostro voto è favorevole per il lavoro fatto, per l'attenzione del Governo il quale, con spirito di cambiamento,

con un decretino - come l'abbiamo definito - che trattava completamente altro e che, rispetto ai grandi temi della ricostruzione, incideva solo per un centesimo - pur importante, evidentemente

del relatore), alla doppia difformità, alla vicenda definita giornalisticamente di nonna Peppina, e via dicendo. Ma la cosa che reputo maggiormente interessante e su cui mi voglio concentrare è

Noi abbiamo un pericolosissimo collo di bottiglia negli uffici speciali per la ricostruzione, negli USR regionali, determinato dalla carenza di personale, dal fatto Se, tra qualche giorno, la ricostruzione ripartirà - e probabilmente ripartirà anche grazie alle cose positive di questo decreto-legge - si fermerà immediatamente, perché negli uffici regionali non ci sono persone che vi lavorano. Le pratiche saranno ammucchiate sopra le scrivanie e resteranno lì; creeranno muri di arretrato che i cittadini continueranno a sollecitare. Ci troveremo davanti a una grande massa di problemi determinati dai ritardi delle pratiche.

relative a questa disparità normativa, che creano problemi seri nella ricostruzione, che andavano affrontate e andranno affrontate rapidamente e

Al di là dell'avvalorare la buona volontà e la consapevolezza da parte di tutti noi di aver fatto emergere la situazione del cratere,

delle coperture; davanti al muro dei Ministeri che spiegano - ma non spiegano - e alle relazioni apodittiche e alle affermazioni che non riusciamo a definire; davanti a tutto

fortemente preoccupati sia per il rischio di ulteriore infrazione rispetto al percorso illustrato dal sottosegretario Castelli, sia per i tempi, perché francamente, se fosse un mille proroghe, non si capisce perché arriva nel

è assolutamente fondamentale per sapere come procedere. La seconda questione è la legge quadro sui disastri naturali. Ne ha parlato il senatore Errani; l'abbiamo detto tutti in sede di Commissione e le audizioni hanno chiarito

il Partito Democratico voterà questo provvedimento (è l'ultimo atto del Governo Gentiloni Silveri, che abbiamo preparato e voluto fortemente) perché è necessario (e lo è per le popolazioni colpite) e ha due ragioni fondamentali: non far venire meno tutte le protezioni sociali per i cittadini che abbiamo costruito in questi mesi; superare gli impedimenti all'*iter* di ricostruzione emersi in corso d'opera solo recentemente. Lo voteremo, ma lo avremmo voluto diverso,

Signor Presidente, la materia di questo decreto-legge non è come le altre. La parola «terremoto» è difficile anche solo da pronunciare senza avvertire una fitta. Penso alla forza, alla dignità, all'esempio di una popolazione colpita ripetutamente da un evento sismico senza precedenti. Migliaia di scosse ancora continuano e hanno spaccato la spina dorsale dell'Italia: l'Appennino centrale, i monti Sibillini, quelli che Leopardi chiamava i monti azzurri; e poi la fascia tra L'Aquila e Rieti, un pezzo di montagne e colline che unisce le Marche, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, comunità di valori che con San Benedetto furono il centro propulsivo della prima costruzione sociale e culturale d'Europa; territori inestimabili, non possiamo perdere; territori bellissimi e difficili che vivono da molto tempo una crisi economica, strutturale e sociale che, dapprima del sisma, mettono a rischio di abbandono e desertificazione, in particolare a danno delle generazioni più giovani. allora niente di più urgente di questo decreto-legge, perché niente è più urgente delle attese e dei bisogni di chi combatte per rialzarsi. La posta in gioco è il nostro destino, la sorte di una parte vitale del Paese.

in alcun frangente, con Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Vasco Errani, Paola De Micheli e tantissimi altri. Abbiamo agito sempre con spirito unitario, cercando la coesione di tutte le forze politiche e il coinvolgimento delle autonomie locali e dei soggetti sociali, mettendo in campo un modello avanzato avanzato che raccoglie le migliori prassi dei terremoti recenti, con l'obiettivo strategico e inderogabile di ricostruire tutto tutto il tessuto urbanistico e comunitario preesistente, con una copertura totale delle spese. Colleghi, le risorse da noi stanziate e che voi - maggioranza e nuovo Governo - avrete il compito di gestire e di non dilapidare

duro, in continua evoluzione, certamente fatto anche di errori, criticità, rigidità e di un'iniziale eccessiva centralizzazione. Ma, di fronte ai problemi, noi abbiamo saputo rimettere in discussione le norme e modificato le cose che non funzionavano, in particolare quando l'*escalation* del sisma ne ha radicalmente cambiato la natura, allargando esponenzialmente il cratere, fatto soprattutto di piccoli Comuni montani e collinari, con moltissime situazioni di dissesto idrogeologico. Il primo nostro impegno è stato proteggere le persone, metterle al riparo e fare scudo dalle difficoltà economiche. Questo è il perno fondamentale di tutto il nostro lavoro degli ultimi due anni, di cui andiamo orgogliosi. Possiamo dire a testa alta che nessuno è stato lasciato solo, con l'integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti; il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli artigiani e alle partite IVA; la sospensione del pagamento di mutui e bollette; i versamenti contributivi e tributari; l'introduzione della busta paga pesante; la cassa in deroga per i lavoratori delle imprese del cratere; il contributo di autonoma sistemazione, che è stato una misura reale di *welfare* a garanzia dei singoli e soprattutto delle famiglie e della loro coesione. ripeto, nessuno - può negare che mai prima d'ora c'era stato un sostegno di questo livello per le necessità economiche della popolazione e la ripresa delle attività produttive. misure legate tra loro, che compongono un progetto, una visione, un'idea di società e un'idea di sviluppo. Se oggi il cratere è vivo - e lo è - è merito di questi strumenti. Signor Presidente,

di cosa significano 600.000 persone colpite e oltre 50.000 sfollati. Eppure, in tutti questi mesi - e ancora adesso - gli sciacalli non si sono fermati, strumentalizzando le difficoltà e seminando sfiducia, zizzania, polemiche e veleni, alimentati ad arte sui *social network* da chi nel cratere probabilmente non ha mai messo piede. Noi siamo orgogliosi di quanto fatto e moltiplicheremo il nostro impegno dall'opposizione, vigilando con il massimo della determinazione affinché non venga vanificato il lavoro indispensabile, fatto tra mille difficoltà, in questi anni. Vigileremo che questo Governo non ci faccia andare indietro, non volti le spalle ai territori e alle popolazioni colpite. Siamo preoccupati, Presidente; preoccupati perché nel cosiddetto contratto - altro non è che un patto di potere tra Salvini e Di Maio su 18.000 parole non ce n'è neanche una su terremoto e ricostruzione. Su 18.000 neanche una parola! Questo è gravissimo. Dite al presidente Conte - che oggi non è qui - che non basta farsi vedere qualche ora, in fretta e furia, nelle zone terremotate, se non si ha un'idea di ciò che bisogna fare. Siamo preoccupati, perché alla gran parte delle nostre proposte, per continuare a sostenere redditi, lavoratori, cittadini, imprese, sindaci, soprattutto quelli dei piccoli Comuni, voi avete detto no. Voi dite di non avere soldi per i terremotati,

Avete detto no a dilazionare i pagamenti sospesi fino a 120 rate; no alla riduzione al 40 per cento dell'importo da restituire; no all'estensione della proroga dell'*una tantum* di 5.000 euro per i professionisti e per le partite IVA; no alla proroga della zona franca urbana per le imprese; tutte misure inserite da noi e che voi adesso state togliendo. Avete detto no alla destinazione del 4 per cento del fondo complessivo per la ricostruzione allo sviluppo economico e sociale dei Comuni del sisma; no all'incremento delle risorse per il servizio civile, per i giovani del cratere; no a tutto quello che riguarda le risorse umane, il personale, anche la polizia locale. Interromperete rapporti di lavoro indispensabili per le esigenze delle aree del sisma. Non sono no al PD: sono no a istanze reali, sentite, chieste a gran voce dalle forze sociali, economiche, professionali. Avete detto no, eppure in campagna elettorale queste cose le avevate promesse. Avete preso i voti e siete scappati.

e ne siamo lieti - tutti sono confluiti: un sì che dà certezza a oltre 500 lavoratori della Whirlpool di Comunanza e alle loro famiglie; un'azienda strategica per il futuro manifatturiero di quei territori, che fa da traino a un indotto numerosissimo. Un emendamento porta questa vertenza in Parlamento ed è una prima vittoria. Adesso toccherà al Governo reclamare un rilancio industriale del sito produttivo, che oggi è pesantemente a rischio. C'è il rischio di 131 esuberi, una vertenza che non ha carattere locale, Presidente, ma che è emblematica di come noi intendiamo la sfida della ricostruzione. Non basterà, infatti, ricostruire solamente i muri; servono una progettualità specifica, un rilancio strategico, ben oltre la proroga dello stato di emergenza. Chiediamo investimenti, anche europei, fuori dal patto di stabilità, per un nuovo modello di sviluppo delle fasce appenniniche, per un *welfare* sanitario e formativo *ad hoc* per quelle zone, per i loro distretti agroalimentari, zootecnici e artigianali, che in un unico piano possono moltiplicare le loro potenzialità. Signor Presidente, serve legare in un'unica vertenza presente e futuro, perché non c'è l'uno senza l'altro. Per qualcuno il terremoto è un evento lontano; non per noi. Per qualcuno sono immagini sbiadite; non per noi. Per noi è e sarà una questione nazionale dirimente e la faremo valere sempre.

a quasi due anni di distanza dall'inizio degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, con 299 morti e oltre 50.000 persone assistite, l'emergenza non è terminata, mentre la ricostruzione è ancora al palo. sono le problematiche che si sono verificate, soprattutto quelle di natura procedurale. La Lega lo avevo detto da subito: è sbagliato prendere una legge, quella del terremoto dell'Emilia, che già allora aveva dimostrato i suoi limiti

troppe le ordinanze (anche qui 59), spesso in contraddizione; tante le incertezze che rallentano la ricostruzione e a soffrire sono i cittadini, migliaia dei quali, sradicati, sono stati costretti a spostarsi in località lontane, in attesa delle SAE, promesse da Renzi in sei mesi,

A soffrire sono anche le imprese. Chi ha mantenuto con coraggio le attività sta subendo un netto calo del fatturato per lo spopolamento da parte dei residenti e per la riduzione del turismo. Mi fanno sorridere i colleghi del Partito Democratico quando nei loro interventi in Aula e alla stampa, accusando questa maggioranza, cianciano di disarmante minimalismo e di pochezza di interventi. Ma, scusate: vi è noto che prima di questo decreto-legge gli ultimi due Governi di Renzi e Gentiloni Silveri per questo terremoto sono intervenuti con otto provvedimenti successivi? Questo decreto-legge era stato annunciato come un provvedimento corposo. Invece, l'Esecutivo Gentiloni Silveri ha varato un mini decreto, un decretino *(Applausi dai Gruppi L-SP e M5S)*. Questa maggioranza, avendo ben presente le esigenze delle comunità colpite, i drammi di famiglie e imprese che hanno perso tutto, anche la speranza, ha fatto una scelta politica responsabile e coraggiosa. Considerando i tempi limitati a disposizione e un bilancio dello Stato blindato, visto che le risorse sono già state allocate da voi del Partito Democratico, abbiamo voluto comunque ampliare la portata del provvedimento. Abbiamo fatto un ciclo di audizioni. Poi, con la fase emendativa, abbiamo introdotto con il contributo di tutti misure fiscali, ma soprattutto inserito anche diverse norme urbanistiche mirate a velocizzare la ricostruzione. Altro che non c'è nulla nel provvedimento, caro collega Saccone di Forza Italia! Sono tante le novità introdotte con il contributo di tutti. Abbiamo prorogato lo stato di emergenza. Abbiamo prorogato la restituzione dei mutui dei Comuni. Abbiamo esonerato i Comuni dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata. Abbiamo prorogato di due anni i mutui per attività economiche e privati per la prima casa. Abbiamo riconosciuto ai privati le spese per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per il cantiere di ricostruzione. Abbiamo prorogato sino al 2020 l'esenzione delle bollette delle forniture in zona rossa, importante per le imprese. Abbiamo aumentato la soglia dell'importo lavori pubblici per l'obbligatorietà della SOA, di cui molte imprese edili locali sono sprovviste. Ciò limiterà l'esclusione dalle gare evitando ulteriori fallimenti. Abbiamo introdotto il rimborso delle spese per l'adeguamento antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo ampliato le centrali uniche di committenza per superare una limitazione eccessiva per i soggetti attuatori. Sono stati prorogati a fine dicembre gli interventi di immediata esecuzione e presentazione delle schede Aedes da parte dei professionisti. Abbiamo previsto la realizzazione di aree turistiche attrezzate per *roulotte* e

di linee guida del commissario con procedure e adempimenti connessi alla costruzione. Per nonna Peppina abbiamo introdotto finalmente una norma adeguata a sanare le casette temporanee costruite senza permesso in emergenza,

ad altre situazioni analoghe, una sanatoria ma a precise condizioni ed è incredibile che sul punto ci siano stati i parlamentari del Partito Democratico che hanno dato dal ciarlatano a Salvini e alla Lega, prendendosi un merito che non hanno

Era della Lega l'emendamento che il Governo PD ha recepito nell'ultima legge di bilancio 2017, ma modificandolo e riducendone drasticamente la portata, tanto che solo nonna Peppina e pochissimi altri, a distanza di mesi e producendo quintali di carte bollate, forse riusciranno a ottenere il dissequestro della casetta e a sanare la situazione. Noi qui abbiamo voluto pensare anche agli altri. Altre modifiche: abbiamo introdotto una norma per consentire demolizione e ricostruzione di abitazioni inagibili in deroga al vincolo stradale. Abbiamo introdotto la possibilità per le diocesi di intervenire su gran parte delle 3.000 chiese danneggiate, ricorrendo a procedure più rapide e - molto importante - per sbloccare la ricostruzione dei privati abbiamo definito le procedure sia per condoni pendenti, sia per sanare le piccole difformità connesse a fabbricati danneggiati dal sisma, e tanto altro ancora. Abbiamo dato risposta a tutte le richieste delle comunità terremotate? No. Mettiamo naturalmente in conto che potranno arrivare critiche da cittadini, imprese, professionisti e tanti altri come i sindaci, che da troppo tempo vivono in uno stato di abbandono, di incertezza per il futuro. A loro, però, assicuriamo che che in queste condizioni abbiamo fatto il massimo in questo decreto-legge, mettendo il massimo impegno. M5S);*impegno che non termina qui oggi. Molte misure saranno introdotte con la prossima legge di bilancio o in un provvedimento dedicato che si occuperà non solo delle problematiche del terremoto del Centro Italia, ma anche di quelle ancora aperte del terremoto dell'Emilia-Romagna

Quello che come Lega però riteniamo inaccettabile è che ci siano esponenti del Partito Democratico che, dopo due anni, si svegliano dal letargo e ora vengono a farci la lezioncina,... *(Applausi

Altro che aspettare Lega e MoVimento 5 Stelle alla prova dei fatti: sono i terremotati che hanno aspettato inutilmente due anni. Voi siete ridicoli. e FI-BP)*. Mi avvio alle conclusioni ringraziando il commissario De Micheli per la correttezza istituzionale avuta; gli uffici della Commissione speciale; il relatore collega Stefano Patuanelli e, in rappresentanza di tutti i componenti della Commissione, la Presidente facente funzioni Erica Rivolta per la grande mole di lavoro svolta in pochissimi giorni. e M5S)*. Gratitudine a oltranza rivolgiamo anche a chi sta operando da due anni nei territori colpiti: i rappresentanti dei Vigili del fuoco, la Protezione civile, L-SP e M5S)*, le diverse organizzazioni di volontariato, i professionisti volontari che stanno aspettando da anni le spese sostenute, i sindaci e gli amministratori comunali. Come maggioranza e come Governo che il terremoto lo hanno inserito nel contratto di Governo, caro collega Verducci, ci mobiliteremo per una ricognizione seria di tutte le criticità, affinché possano essere superate. Valuteremo la necessità di una legge-quadro, un quadro normativo unico che superi le frammentazioni e le contraddizioni legislative. Ma, soprattutto, ci impegneremo per mettere in atto un piano di ricostruzione strategico di prevenzione e salvaguardia del territorio che rilanci socialmente ed economicamente le zone colpite in grado di rappresentare anche un fattore di sviluppo dell'intero Paese. Il Gruppo Lega-Salvini Premier voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

questo problema è stato sollevato anche dalla commissaria in sede di audizione e c'è un documento scritto

degli aiuti, che è una responsabilità di questo Governo. Non ha risolto, perché non ha voluto vedere quello che è stato fatto dai Governi di centrodestra, la questione fiscale, giustamente ricordata dal collega Pagano, per cui si poteva tranquillamente arrivare a una riduzione dell'IRPEF al 70 per cento e a una rateizzazione a 120 rate, fatta dal nostro Governo nel 2009 e non riconfermata, ovviamente,

terremoto dimenticato. Allo stesso modo, come ha detto qualche altro collega, c'era il problema dell'Emilia e della Lombardia. Il grumo della non attenta gestione delle risorse si si è poi riverberato sul sostegno al reddito, perché deve essere chiaro, in quest'Assemblea, che le misure di sostegno al reddito sono state praticamente scaricate sui bilanci delle Regioni: non è stato fatto niente

agenti di polizia municipale - checché ne dica il relatore - perché non è stato approvato l'emendamento a firma Gasparri-Mallegni nel merito.

quello che era stato detto in audizione. Non c'è una targa su quegli emendamenti, perché è un lavoro di Commissione, e ve lo abbiamo anche detto: non è corretto!

quelle norme che ci avevano suggerito i tecnici della Protezione civile, noi le abbiamo tradotte in emendamenti che poi sono stati assorbiti. Quindi, non è che è stato fatto qualcosa da qualcuno: è stato fatto qualcosa tutti insieme, un grande pezzo è rimasto il motivo per cui noi riteniamo che si debba esprimere un voto di astensione è perché il pezzo che è rimasto fuori è importantissimo Noi abbiamo predisposto emendamenti di tutti i generi, che abbiamo presentato e sono agli atti. Forza Italia si è impegnata perché, giustamente, ha preso l'impegno

il decreto-legge è stato emanato per evitare la scadenza di norme a favore delle popolazioni colpite dal sisma e, riassumendo brevemente, contiene: la proroga delle scadenze della busta paga pesante; la proroga e sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi; la sospensione del pagamento del canone RAI e delle principali utenze domestiche; la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018 con la possibilità di estensione di ulteriori dodici mesi; un emendamento per regolarizzare le tante casette di legno abusive costruite in via autonoma dagli sfollati,

possibilità per i Comuni di realizzare delle aree attrezzate e tanti altri interventi. Alcuni numeri: 300 milioni per la proroga dello stato di emergenza; 10 milioni per consentire la costruzione di attrezzature e aree turistiche per *camper* e *roulotte* per possessori di seconde case. Abbiamo Abbiamo dato la possibilità di spalmare, a partire dal primo gennaio 2019, i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro. Ci sono 700 unità di personale che stanno lavorando nei 130 Comuni. L'ANCI e Forza Italia richiedevano una ulteriore proroga oltre il 31 dicembre del 2018, ma per questo provvedimento si rimanda alla legge di bilancio del prossimo autunno, nella quale c'è la volontà di stanziare risorse apposite. Per tutte queste cifre sono state individuate le relative coperture finanziarie. Ci preme sottolineare come, per intervenire sulle lievi difformità, in sede di Commissione speciale non sia stata data mano libera ad alcun abuso. Il Movimento, sin dalle sue origini, ha sempre condannato abusi e condoni. Quello che è stato inserito è la possibilità di costruire per modifiche non strutturali, come dovrà essere accertato dai tecnici professionisti. Nel decreto è anche inserita la proroga per i primi sei mesi del 2019 della cassa integrazione in deroga per lo stabilimento Whirlpool. Non abbiamo avuto difficoltà a sostenere questa parte del decreto-legge, anche se il primo firmatario è stato il Partito Democratico. I colleghi dell'opposizione sanno bene che la questione della perdita del lavoro e e non solo dei lavoratori della Whirlpool sta a cuore a tutto il Movimento: a noi non interessa chi presenta un emendamento, a noi interessa il bene del Paese! Il ministro Luigi Di Maio ha fissato un tavolo tecnico per il 6 luglio, nel quale si incontreranno proprietà e parti sociali per dare garanzie occupazionali e non solo sussidi in eterno. Si evidenzia inoltre come questa crisi sia l'ennesima a cui assistiamo nel Paese, a seguito di una politica industriale dissennata, operata

e si sono persi 1.500 posti di lavoro e molti di questi non sono stati persi nell'area del cratere. Le opposizioni diranno che si tratta della crisi economica, ma, come è stato ribadito anche in Aula, la crisi consiste nell'aumento della forbice, che vede un aumento della ricchezza nelle mani di pochi e la perdita del potere d'acquisto per la maggior parte dei cittadini. È una crisi dovuta a questo modello di sviluppo socioeconomico, voluto dai Governi che ci hanno preceduto! Le opposizioni e in particolare il PD hanno posto l'accento sul fatto che ci siano stati vari emendamenti tagliati. È il gioco della politica presentare emendamenti per poi dire che il Governo non ha risposto a delle sacrosante richieste del Paese con estrema ipocrisia. Ricordo che il Governo ha dato 20 miliardi di euro ai banchieri e nell'area del terremoto sono state

Il provvedimento è stato emanato pochi giorni prima della scadenza e il Governo ha dovuto intervenire immediatamente dopo l'insediamento, dunque con tempi estremamente ridotti. Le richieste principali dei cittadini colpiti, nei limiti consentiti dalla legge e delle coperture finanziarie, sono state realizzate. Il tema della vulnerabilità sismica delle scuole non ha certamente avuto il giusto risalto: si tratta purtroppo di un grave problema, comune a tutto il Paese. Si ricorda, però (in particolare ad uno smemorato PD), come la regia degli interventi sia stata in mano loro per due anni. Il senatore Verducci parla di modello di intervento avanzato, ma non si chiede come mai, a distanza di due anni, tutta la ricostruzione deve ancora partire. Non ha letto bene il contratto di Governo, che cita testualmente. Le decisioni devono essere assunte con cognizione di causa ed appare evidente anche all'ultimo scolaretto che il Governo non può prendere decisioni se prima non ha valutato la situazione socioeconomica: quella situazione che però era ben nota a chi ha governato da anni e aveva in mano tutti i documenti necessari a prendere le decisioni e si è accorto che c'erano miglioramenti da fare solo dopo che il decreto emanato dalla propria commissaria era stato presentato. Per tale motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento in

Colleghi, se dovessimo stabilire un applausometro, dovrei dire che questa è la legislatura dei *record* che non si sono mai verificati.

di parlare il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Di Maio. [DI

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicarmi e che vorrete dedicare a questa informativa su un tema importantissimo, che è quello degli infortuni sul luogo di lavoro. È un tema su cui stiamo lavorando come Governo e che parte da dati che sono molto preoccupanti. I lavoratori continuano a cadere come soldati sul campo di battaglia. Pochi giorni fa a perdere la vita è stato un operaio veneto, che voglio ricordare in quest'Aula, Pasquale Misitano, di 42 anni, l'ultima delle oltre 300 vittime di infortuni sul lavoro dall'inizio di quest'anno. Pasquale lascia una moglie, due figli e un terzo in arrivo che purtroppo non conoscerà mai. Un profondo cordoglio e la vicinanza vanno ai suoi parenti e a tutte le famiglie dei lavoratori vittime degli infortuni mortali, e a tutti quei lavoratori che nella loro vita professionale hanno subito infortuni gravi e invalidanti.

I numeri che vengono dall'INAIL sono devastanti e assomigliano a un bollettino di guerra, per quanto mi riguarda. Nei primi quattro mesi del 2018 sono stati 286 i lavoratori morti sul lavoro, con un incremento del 9,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. I morti oggi sarebbero 349: una media di 2 persone ogni giorno e purtroppo il dato reale potrebbe essere addirittura più alto, considerando i lavoratori non tutelati dall'INAIL e le denunce di infortunio mortale non riconosciute come tali dall'INAIL, a tutto il mondo del lavoro in nero. L'elenco delle persone che perdono la vita mentre svolgono il proprio lavoro purtroppo si allunga ogni giorno. Prima della persona che ho ricordato all'inizio del mio discorso, hanno trovato la morte Salvatore Lombardo, operaio nello stabilimento Fincantieri, di 43 anni; Davide Olivieri, che è morto a soli 22 anni, schiacciato da un muletto; Giuseppe Cicero, che a cinquant'anni ha perso la vita travolto dal suo trattore; Biagio Amendolia, di 63 anni, caduto da un'impalcatura. Lasciatemi dire che se la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere prima di tutto una cultura, questa cultura della sicurezza la devono avere in primo luogo gli edifici pubblici dello Stato e le aziende partecipate dello Stato. Queste morti vengono definite «morti bianche» e in realtà molto spesso non hanno nulla di candido, ma derivano dalla trasgressione delle norme basilari di sicurezza. Il *trend* dei primi cinque mesi del 2018, come detto, registra un aumento degli infortuni, ascrivibili principalmente a cadute dall'alto, a investimenti a opera di mezzi o macchine, a intossicazione in ambienti confinati, a ribaltamento di mezzi meccanici specialmente in agricoltura. Tra gennaio e dicembre 2017 le denunce di infortuni pervenute all'INAIL sono state 635.433, in linea con quelle rilevate nell'analogo periodo del 2016. La diminuzione di 1.379 casi (pari a -0,2 per cento) è dovuta al calo degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, mentre quelli *in itinere* nel tragitto casa-lavoro e viceversa hanno avuto un incremento pari al 2,8 per cento. Voglio essere molto chiaro qui, da Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ma anche da Ministro dello sviluppo economico: non sono uno di quelli che pensa che la sicurezza sul lavoro si possa ottenere esclusivamente scaricando sulle imprese oneri e responsabilità, ovvero attraverso l'esclusivo uso di misure punitive nei confronti delle imprese e degli imprenditori. C'è bisogno di sensibilizzare datori e dipendenti verso una cultura della sicurezza del rischio, attraverso attività di informazione e formazione. Sicuramente bisogna rafforzare le attività ispettive di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative competenti, ma quando queste strutture

aziendali e premiare le imprese che investono nella sicurezza, puntando sulle agevolazioni. Dobbiamo ridurre i costi, agevolando il valore dell'IVA sugli acquisti effettuati dai datori di lavoro per quanto riguarda i prodotti relativi alla sicurezza per le aziende. In generale, ci tengo a trasmettere a quest'Assemblea una mia convinzione, maturata negli anni in cui sono stato parlamentare. Non è con più leggi e ancora più leggi che otterremo il risultato di tutelare i lavoratori. consegue proprio andando nella direzione opposta, che è quella di cominciare ad attuare e far rispettare le leggi esistenti e, con meccanismi premiali, iniziare a premiare chi non solo rispetta le norme, ma fa anche meglio di quello che la legge sulla sicurezza sul lavoro Dobbiamo potenziare di più i controlli, lo abbiamo detto, ma, allo stesso tempo, ridurre la burocrazia a favore di chi vuole rispettare le norme contro gli infortuni sul lavoro, che non può essere obbligato a compilare decine e decine di scartoffie per mettersi in regola. Questo concetto non vale solo per la tutela lavorativa per chi ha già diritto alla tutela INAIL. Gentili sentori, c'è tutta un'altra categoria, ci sono tante altre persone, tanti altri lavoratori che, visto il mutato nuovo contesto del mondo del lavoro, hanno bisogno di una protezione sociale e non ce l'hanno. Come primo atto da Ministro del lavoro ho deciso di aprire le porte del Ministero del lavoro ai cosiddetti *riders*, nuove categorie lavorative che fanno parte di nuovi tipi di economia. Li ho coinvolti direttamente, ho ascoltato le loro voci e aperto un dialogo per pianificare un tavolo tra queste grandi compagnie della cosiddetta *gig economy*. Questi ragazzi, che consegnano pietanze in bici utilizzando una App e che spesso non hanno neanche un contratto (figuriamoci una tutela), sono stati i primi lavoratori a entrare al Ministero del lavoro di questo Governo. È nostra intenzione cominciare a introdurre una tutela per queste categorie, anche collaborando con le aziende.

al Consiglio europeo dei Ministri del lavoro abbiamo provato a inserire in una delle direttive che si stava discutendo il concetto di lavoratore, ossia chi è il lavoratore oggi. Infatti, non è detto che

pretendono tutele. Il concetto di chi è il lavoratore e qual è il minimo di dignità che bisogna corrispondere a chi lavora sarà uno di quelli che avremo più a cuore come Governo del Paese.

è andato bene: c'è stata una disponibilità ad aprire il tavolo. Lo dico chiaramente: se ci sarà la disponibilità a dare tutele a questi ragazzi attraverso una concertazione, benissimo. Il Ministero patrocinerà questa concertazione e porterà l'obiettivo di dare tutele ai *riders.* non ci sarà, perché non ci sarà la volontà da parte di queste compagnie di smetterla di sfruttare i nostri ragazzi, allora faremo una norma per tutelarli. *(Applausi Credo che non sia alimentando il conflitto tra datore e dipendente che riusciremo a portare avanti il tema dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo delle imprese. È il momento di fare squadra.

di comune accordo tra proprietà e lavoratori, ci siamo detti: va bene, qui abbiamo giocato in difesa e abbiamo scongiurato la cassa integrazione, con i contratti di solidarietà, ma ora attraversiamo la strada, andiamo al Ministero dello sviluppo economico e investiamo in nuovi modelli di sviluppo, per rilanciare questi settori e non affrontarli sempre con la paura che si stiano perdendo posti di lavoro o che si debba finire in cassa integrazione. La convinzione che datore e dipendente debbano fare gioco di squadra d'ora in poi viene anche da un concetto, quello del *made in Italy* nel mondo. Il *made in Italy* è diventato il nostro ambasciatore ed è stato il nostro ambasciatore più importante nel mondo, anche nei momenti più bui per la reputazione di questa Nazione *(Commenti della chi era imprenditore era sempre anche lavoratore (lavorava nell'azienda) e chi era lavoratore si è sempre sentito anche un po' imprenditore nella piccola e media impresa italiana e ha portato i prodotti più belli e più di qualità che sono sul mercato in giro per il mondo. Porterò avanti questa convinzione nella direzione del Ministero del lavoro e dello sviluppo economico. Tutti i lavoratori, come dice l'articolo 38 della Costituzione, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, che siano questi subordinati o meno, devono avere gli stessi livelli di tutela in caso di infortunio e di malattia professionale da parte dell'INAIL. Il nostro obiettivo è il miglioramento assoluto delle condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Affinché questa azione sia efficace, continuerò a incontrare e a confrontarmi con tutti coloro che rappresentano questo settore. Il dialogo tra le parti è fondamentale e voglio dire chiaramente a tutti i soggetti coinvolti in questo tema che le porte del Ministero - e ci mancherebbe altro - saranno sempre aperte e anche quando non saremo d'accordo, continueremo a confrontarci ad oltranza per trovare una soluzione comune, che riesca a soddisfare il più possibile le parti più deboli della nostra società. Un primo strumento da valorizzare è il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che fornisce dati per orientare, programmare e valutare l'efficacia di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento di questo sistema vede coinvolti, oltre ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche i rappresentanti delle altre amministrazioni competenti, quali i Ministeri della salute, della pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché, ovviamente, l'INAIL. L'effettivo avvio del tavolo tecnico ci consentirà di verificare l'adeguatezza delle modalità di funzionamento del cosiddetto SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza. Un altro tema riguarda gli incentivi economici. Sempre maggiore importanza dovrà, quindi, avere il sistema di informazione e formazione, vero fulcro del sistema preventivo dei rischi e dovremo favorire - l'ho già detto e lo ripeto un sistema di premialità nei confronti delle imprese che decidono di investire sulla sicurezza, di migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro e di impegnarsi nella formazione. È molto importante la collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per instaurare una cultura della sicurezza sul lavoro già dalla scuola potenziando gli strumenti di alternanza scuola-lavoro. va potenziata la ricerca per individuare soluzioni innovative in grado di assicurare a tutti i lavoratori una tutela 4.0. Enti come l'INAIL o in altri Paesi del mondo sono le principali fonti di *venture capital* per le *start-up* innovative. La nostra idea è quella di creare un fondo per le *start-up* innovative cui possano contribuire anche soggetti come

presentazione della relazione del presidente dell'INAIL - l'INAIL pubblicherà un bando per 4,5 milioni di euro concernente tre rilevanti ambiti istituzionali: il reinserimento lavorativo, la tutela assicurativa e la prevenzione. Per il capitolo della vigilanza sui controlli va ricordato che l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene svolta prioritariamente dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio. Però, bisogna mettere le ASL nelle condizioni di fare tutti i controlli con i mezzi adeguati. Solo in alcuni settori di attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, questa vigilanza può essere esercitata anche da uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà molto importante il coordinamento tra gli enti perché la competenza, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, è stratificata; riguarda diversi livelli dello Stato, diversi ambiti territoriali e nazionali alla presentazione della relazione dell'INAIL, io mi impegno a cercare di coordinare il più possibile questi enti, non con leggi impositive che dicano: «Dovete coordinarvi» di quelle ne abbiamo a decine e purtroppo, comunque, non si coordinano ma cercando di favorire la relazione umana di chi ha le responsabilità di questi enti e cercando di favorire un coordinamento politico di queste persone con un Ministro che li metta intorno a un tavolo non solo dia loro degli obiettivi, ma recepisca tutti i *feedback* e tutte le istanze che vengono da questi mondi. Ci tengo qui a evidenziare l'encomiabile lavoro dall'Ispettorato. I 280 ispettori impiegati nell'attività di prevenzione hanno effettuato solo nel 2017 23.000 accertamenti. Per quanto riguarda il tasso di irregolarità delle aziende ispezionate, si è registrato un aumento nel corso del 2017 di circa 3,5 punti percentuali rispetto al 2016, cioè pari a circa il 77 per cento rispetto al 73 per cento dell'anno precedente. Il potenziamento di questi organi ispettivi, siccome le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sostanzialmente limitate al settore dell'edilizia, è possibile attraverso l'emanazione di un atto di alta amministrazione a legislazione vigente, che però dovrà necessariamente essere accompagnato da un incremento del numero delle unità, che oggi non è superiore a 280, un numero non sufficiente. L'Ispettorato ha carenze di organico dovute al cosiddetto blocco del *turnover* e nei prossimi cinque anni il personale ispettivo e non ispettivo subirà quasi un dimezzamento in ragione dei pensionamenti. se vogliamo veramente potenziare l'attività di vigilanza, si dovrebbe prevedere l'assunzione di almeno 1.000 unità, e siamo al lavoro su questo *dossier* dal primo giorno. Se è vero che l'Ispettorato ha avviato un reclutamento di 150 unità, dato non ancora effettivo visto il completamento dei concorsi, questo numero non può di certo colmare le carenze di organico che si sono verificate negli ultimi anni e che si verificheranno nei prossimi anni. Dovremo fare molto di più. C'è anche il tema della disparità tra settori. Ci sono comparti, ad esempio la pubblica sicurezza, le cui norme interne sulla sicurezza sono ferme a vent'anni fa. Serve dar vita al gestore unico delle informazioni sulla sicurezza sul lavoro, fondamentale per prevenire l'infortunio e non intervenire quando ormai è troppo tardi. Un altro aspetto da sottolineare, Presidente, riguarda il ricatto occupazionale:

È fondamentale scardinare la logica del massimo ribasso che governa l'affidamento dei lavori sia pubblici sia privati *(Applausi dai Gruppi questi lavori rientrano nel sistema del subappalto, situazione, questa, nella quale azienda e lavoratore non hanno tempo e modo di seguire un'adeguata formazione. Per non parlare dell'avvalimento, che è un altro di quegli strumenti che fa parte delle normative che vogliamo cambiare. Se vogliamo intervenire, permettendo a chi lavora di scegliersi un lavoro dignitoso, dobbiamo porre in essere uno strumento che esiste in tutti i Paesi europei, la *flexicurity*,

normative. Dobbiamo lavorare alla cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, cominciando, come dicevo all'inizio, dagli edifici pubblici, dai luoghi di lavoro pubblico e dalle nostre partecipate di Stato, perché su questo lo Stato deve dare l'esempio e vedrete come tanti cittadini crederanno molto di più nelle leggi emanate in questi anni sulla sicurezza sul lavoro. L'azione di questo Governo sarà volta non solo a favorire la creazione di nuovi e stabili posti di lavoro al posto del precariato ma anche tutti coloro che lavorano in condizioni di totale insicurezza e che, oltre al lavoro, rischiano di perdere addirittura la propria vita grazie.

UV))*. Signor Presidente, signor Ministro, l'impegno contro le morti sul lavoro non ha colore politico. È grave che, in un Paese avanzato come l'Italia, se ne registrino così tante. Siamo contenti che sia un'informativa su questo tema a inaugurare la sua presenza come Ministro in quest'Aula. Qualcuno parla di bollettino di guerra, le morti bianche vanno a braccetto con la crisi economica e con il fatto che molte aziende hanno ridotto le spese in sicurezza dei luoghi di lavoro. Per questo si devono premiare con incentivi e sgravi fiscali quelle aziende che costruiscono le condizioni ottimali per l'incolumità dei lavoratori, che non sono solo quelle previste dalle norme ma costituiscono un impegno sostanziale, un atto di cura nei confronti dei lavoratori. Lo stesso devono fare i cittadini attraverso i loro comportamenti d'acquisto. Così come c'è una sempre maggiore attenzione verso quelle imprese che producono secondo principi etici di sostenibilità ambientale, i consumatori devono porre la stessa attenzione sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza. Insomma, ministro Di Maio, credo ci siano tanti margini di miglioramento dal punto di vista normativo e della sensibilità pubblica per contrastare il fenomeno.

soprattutto quelle agricole. Per queste imprese di ridotta dimensione e a conduzione perlopiù familiare, l'introduzione di nuove norme non ha portato a un miglioramento delle condizioni di sicurezza per la relativa semplicità del processo lavorativo e per il basso rischio dei macchinari adoperati. La burocrazia per aziende così piccole è un freno alla produzione e un disincentivo a continuare l'attività e questo in montagna è un problema anche per la tenuta del tessuto sociale e per la funzione di presidio del territorio per il contrasto al dissesto idrogeologico. È solo un esempio ed altri se ne potrebbero fare. Pertanto, signor Ministro, va bene operare per combattere questa piaga delle morti sul lavoro, ma facciamo in modo che le misure aggrediscano davvero il problema da cui origina il rischio. quindi con decisione, ma con grande attenzione, valutando attentamente tutti gli aspetti. Signor Presidente, Signor Ministro, è impossibile, oltre che poco dignitoso, racchiudere in cinque minuti una discussione e una riflessione su un tema drammaticamente complesso come quello della sicurezza sul lavoro.

È una fredda contabilità, dietro alla quale poi si nascondono storie di lavoratori gravemente feriti proprio nel luogo in cui avrebbero dovuto sentirsi più protetti, cioè il proprio posto di lavoro, oppure storie di vite drammaticamente spezzate. Le proposte sono quelle che ho ascoltato anche in quest'Aula: lavorare sulla cultura della prevenzione, coinvolgendo sindacati e imprese; utilizzare i processi di automazione e innovazione tecnologica, proprio per svolgere i lavori più pericolosi; aumentare significativamente il numero degli ispettori sul lavoro. Va bene infatti il meccanismo premiale, ma se qualcuno non rispetta le regole è giusto che sia sanzionato e punito. Penso che si debba fare questo. Naturalmente anche le misure di defiscalizzazione degli investimenti per le spese che riguardano la sicurezza vanno bene e il Governo, se si avvierà velocemente nella direzione di misure di questo genere, troverà il nostro consenso. Dobbiamo però essere consapevoli di un punto: non si può affrontare il tema della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e sul lavoro senza capire bene qual è il modello di organizzazione del lavoro - e, vorrei dire, dei sistemi di produzione - che si sta imponendo nel tempo che viviamo. L'ha detto in qualche modo anche lei, signor Ministro: c'è un nesso stringente tra i morti che piangiamo quotidianamente, questa triste contabilità, e il fatto che si stanno imponendo un modello e un meccanismo per cui l'aleatorietà

avvenendo nel meccanismo del massimo ribasso, quando c'entra il pubblico, e anche in quello della catena di appalti e subappalti, in cui si perde di vista la titolarità delle responsabilità anche in relazione al tema della sicurezza sul lavoro. Non si capisce più chi è responsabile e i fenomeni del lavoro nero arrivano anche da quel tipo di condizione e di contesto. Per questo penso che si debba partire da questa riflessione più larga e organica,

e, ad esempio, per i lavoratori in un settore delicatissimo, perfino infiltrato dalla criminalità, come la logistica, e per i milioni di lavoratrici e lavoratori nei settori più disparati di questo Paese. Glielo dico, signor Ministro, cercando di darle un consiglio con il massimo rispetto: la smetta di sfarfalleggiare da un tema all'altro inseguendo la moda del momento.

basta inseguire iniziative che si consumano nello spazio di una conferenza stampa o in un *live* su Facebook, cosa di cui lei è maestro. Bisogna affrontare il lavoro nella sua complessità

è dal 1955 che questo Paese non istituisce presso le più alte istituzioni dello Stato una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla condizione dei lavoratori; era

nella realtà del lavoro di questo Paese e di che cosa è diventato. Abbiamo bisogno che lo si capisca anche attraverso uno strumento come quello di una Commissione d'inchiesta che ha poteri paragonabili a quelli della magistratura, perché anche così si affrontano i temi della sicurezza sul lavoro. Se infatti non si deve morire di lavoro, come consiglierebbe la saggezza di una società moderna, visto che semmai dovremmo liberare le donne e gli uomini dal tempo

Signor Ministro, quante volte ognuno di noi ha letto o sentito dire: «È stata una disgrazia» oppure: «È successo l'imprevedibile» o, ancora, «Eppure per quarant'anni aveva svolto quella mansione senza mai un problema»?

Guardate, nessuna speculazione politica su un argomento così importante e delicato; non voglio attribuire responsabilità a questo o a quel Governo; non mi interessa e non interessa a noi del Gruppo Fratelli d'Italia. Ciò che invece ci interessa maggiormente è la realizzazione di un vero ed efficiente piano di sicurezza sul lavoro che passi dalla formazione permanente alla responsabilizzazione delle aziende e dei lavoratori. Non è accettabile che nel 2018 sia ancora possibile morire schiacciati da un trattore o da un muletto, o all'interno di una cisterna o precipitando dal tetto di un capannone. Diciamo basta agli appalti al massimo ribasso, agli infiniti subappalti che di fatto si sostengono propinando condizioni di lavoro paragonabili allo schiavismo. Oggi sono stati citati numeri, gli ennesimi, che ci raccontano di una strage che non finisce mai. Chiediamo al Governo e a lei, signor Ministro, agevolazioni alle aziende per la formazione, per gli investimenti per la sicurezza: prevenire e formare deve essere conveniente e non produrre ulteriore burocrazia.

riguardante il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che è rimasto lettera morta per tutti quei settori ad alto tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti complessità organizzative e da gravi fenomeni di concorrenza sleale. Questo complesso di norme inattuate produce una serie di effetti negativi: assenza di tutela per i lavoratori, profonde incertezze nella gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro. 300 i morti al 14 giugno, cifra che sappiamo inesatta perché altre morti di lavoratori in nero, vittime del caporalato, spesso non vengono conteggiate.

Se anche i 34 casi ancora in istruttoria risultassero tutti riconosciuti sul lavoro, si arriverebbe a 651 morti, con un calo del 2,8 per cento rispetto ai 670 del 2016 (che costituisce il minimo storico dal 1951). Lo si legge nella relazione annuale INAIL. Le denunce di infortunio sono state 641.000, in linea con il 2016, e ne sono state riconosciute sul lavoro 417.000, di cui il 19 per cento fuori dall'azienda.

Purtroppo, nei primi cinque mesi del 2018 sono arrivate all'INAIL 389 denunce di infortunio mortale, con un aumento del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 (14 casi in più). è stato reso noto dalla relazione annuale dall'INAIL, che sottolinea come l'aumento riguardi solo i casi avvenuti *in itinere*, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (passati da 104 a 118), mentre per quelli occorsi «in occasione di lavoro» le denunce sono state 271 in entrambi i periodi. In particolare voglio sottolineare alcune cose che ritengo estremamente rilevanti: sulla base di dati recenti riferiti al 2017 è nel settore dell'edilizia, insieme a quello dell'agricoltura, che si concentra il maggior numero di incidenti sul lavoro; il numero degli infortuni gravi o mortali aumenta considerevolmente, specie se si considera «infortunio sul lavoro» un incidente stradale che vede coinvolte persone negli spostamenti legati all'attività lavorativa; lavorativa; gli autotrasportatori spesso sono vittime di incidenti per il superlavoro, a causa della concorrenza sleale dei camionisti dell'Est che viaggiano senza regole e a prezzi molto più bassi rispetto ai nostri. Per restare competitivi, i nostri devono ammazzarsi di lavoro, spesso anche letteralmente. Per affrontare tale complessa problematica è molto importante implementare l'attività di prevenzione e di sensibilizzazione: sarebbe opportuno istituzionalizzare gli eventi ad essi dedicati, soprattutto nelle scuole, in specie quelle professionali. Signor Ministro, nella sua informativa alla Camera e in numerose altre dichiarazioni pubbliche - tra cui anche quelle di oggi - lei ha preso un impegno solenne: combattere la precarietà (attraverso l'introduzione, in particolare, di una serie di tutele per i *riders*). È una sfida importante per il futuro dei nostri giovani, ma la sollecito a intervenire anche a favore dei tanti ricercatori degli IRCSS, che attendono da decenni la stabilizzazione dei loro contratti. Si tratta di persone altamente qualificate che garantiscono l'attività di studio, ricerca e innovazione nel settore sanitario e che, in mancanza di un'attenzione concreta, sono condannati a emigrare all'estero o a cercare impiego in aziende private. Signor Ministro, concludo con una frase

sua presenza era dedicata esclusivamente e in particolare alla questione riguardante gli incidenti sul lavoro e le cosiddetti morti bianche. Le dico questo perché nelle ultime settimane, all'avvio di questo suo Governo, il Governo del cambiamento, noi abbiamo davvero assistito a un'operazione di distrazione di massa:

signor Ministro, glielo dico proprio con il cuore: ci aiuti a rimettere al centro le questioni cruciali che riguardano il futuro di questo Paese. Il Dicastero che lei presiede è il cuore del Paese. E allora, signor Ministro, vorremmo parlare con lei di Europa, magari riportando all'attenzione di quest'Assemblea i temi indicati dal pilastro europeo dei diritti sociali, che lei ha discusso insieme con noi alla Camera e approvato a Göteborg nello scorso mese di novembre. Parlavamo di una Europa delle pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e dell'investimento in beni comuni pubblici europei: infrastrutture, ricerca, innovazione,

sul reddito di cittadinanza nelle sue numerose variazioni in corso. Ci piacerebbe anche sapere come lei intende riformare la legge Fornero, battaglia del suo Movimento durante la campagna elettorale. Ci piacerebbe sapere come intende modificare la riforma del lavoro. Ci piacerebbe conoscere i suoi orientamenti sui futuri decreti attuativi che riguardano la riforma del terzo settore, che lei non ha votato nella precedente legislatura. Cosa vorrà poi fare del fondo dedicato ai *caregiver* familiari? Come intende muoversi in concerto con il suo collega Ministro senza portafoglio sui temi della famiglia e della disabilità?

la capacità di innovare, garantire sicurezza non soltanto producendo nuovi investimenti in macchinari - pure importanti - ma lavorando in nuove organizzazioni che rendono il lavoratore protagonista.

le chiedo solo una cortesia: non istituisca cabine di regia. La ricordo nei suoi interventi alla Camera dei deputati: quando parlavamo di cabina di regia, diceva sempre che sono una perdita di tempo e che stavamo dilatando i problemi. Se lei vuole affrontare i temi del reddito di cittadinanza e le questioni che ci stanno a cuore e stanno a cuore anche al Partito Democratico, si misuri sulla concretezza e sulle proposte - noi ci siamo e apriremo il confronto - piuttosto che istituire cabine di regia, che danno l'impressione di un ennesimo *escamotage* per rinviare il confronto sulle questioni che riguardano la vita del Paese. La invito ad evitarle: per quanto possibile, riguarda il tema all'ordine del giorno, le ricordo che in Senato una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e, più in generale, sulla sicurezza in ambito lavorativo è stata istituita nella XIV

nella XVII legislatura, ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione molto approfondita, elaborata e propositiva, dalla quale intendiamo riprendere il filo e portarlo lontano.

per quanto ci riguarda, l'impegno rimane fermo e costante. Concludo riprendendo una dichiarazione, penso a lei molto cara, del Presidente della Repubblica - "dimissionato" per alcuni giorni dal suo Movimento - contenuta in un passaggio del discorso del 1° maggio. Diceva il Presidente della Repubblica: «Desta allarme la sequenza - purtroppo continua - degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro. Il nostro pensiero va anzitutto alle vittime, e al profondo dolore dei loro familiari, a cui esprimiamo una sincera

Questi eventi sono causati da circostanze che possono e devono essere evitate. Questo richiama la responsabilità di tutte le parti». Signor Presidente, signor Ministro, noi siamo ancora qui,

drammatica pari a oltre due al giorno. Sono veramente dati e numeri che evidenziano per intero la drammaticità delle morti sul lavoro, che devono quindi essere al centro della nostra attenzione. Noi condividiamo, signor Ministro, le sue considerazioni le sue volontà nell'agire all'interno del Governo per porre un freno a questo dramma. Siamo convinti che l'azione di Governo debba quindi essere indirizzata su due principali rotte, consiste sicuramente in un rafforzamento delle azioni di vigilanza, di controllo e di ispezione, colpendo severamente chi per profitto sfrutta i lavoratori, non rispettando le regole e le norme che in modo consapevole e spregiudicato determinano queste morti. Bisogna colpire severamente coloro che non possono essere definiti imprenditori, non possono essere definiti imprenditori, ma esclusivamente delinquenti che mettono al primo posto il profitto rispetto al compito primario, che è quello di creare sviluppo, occupazione e opportunità. Si tratta però, per quanto riguarda noi, di una minoranza; una minoranza che deve essere colpita e stroncata. È certamente necessario, quindi, rendere più efficace l'azione congiunta delle ASL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro; servono sicuramente più assunzioni, serve fissare delle regole per le quali non possa essere il massimo ribasso il criterio con il quale vengono aggiudicati i lavori pubblici. Tutte queste azioni sono sicuramente necessarie e fondamentali, ma non bastano. Non basta l'azione sanzionatoria. Il problema si risolve non solo con misure punitive, non solo con la repressione, ma soprattutto con la prevenzione. Bisogna aiutare le imprese e gli imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese che ancora oggi, in una fase di piena crisi economica, al di là di quello che vogliono affermare i rappresentanti del precedente Governo, stanno affrontando mille difficoltà, con grande dignità e senso di responsabilità. Questi sono gli imprenditori che vanno tutelati ed aiutati: ogni giorno devono affrontare mille preoccupazioni, mille incombenze, scelte difficili; ogni giorno, quotidianamente. Ci sono troppi costi, troppe tasse, troppi adempimenti burocratici. Questi imprenditori vanno aiutati anche con provvedimenti del Governo, del nostro Governo. Serve dar loro più tempo, più energie e risorse per applicarle alla sicurezza sul lavoro

La nostra analisi rispetto a questi dati ci porta a ritenere che, anche da questo punto di vista, la legge Fornero va cambiata. Non si tratta, quindi, solo di una questione di giustizia sociale: non possiamo essere il Paese che è passato dalle *baby* pensioni all'età pensionabile più alta d'Europa; non si tratta solo di dare più occupazione ai

In definitiva, c'è un altro tema su cui dobbiamo riflettere. Viviamo in una società votata al progresso, che però si misura anche dalla sicurezza sul lavoro, soprattutto dalla sicurezza del lavoro: è una questione vitale e di civiltà. I successi del Governo da cosa verranno misurati? Dal livello dello *spread* o dal rapporto *deficit*-PIL? No, noi non crediamo che questi siano i dati fondamentali su cui verrà misurata da parte dei nostri concittadini l'efficacia dell'azione di questo Governo. Verrà misurata dal livello occupazionale, dal numero di giovani italiani che non emigreranno e che rimarranno a costruire la loro vita e il loro futuro nel nostro Paese. *(Applausi La Lega valuterà i risultati dell'azione di Governo partendo da questi numeri e da questi risultati. Queste sono le priorità del Paese: lavoro e sicurezza sul lavoro. E noi siamo certi che sarete all'altezza di questo difficile compito, vitale per il futuro delle nostre comunità e dei nostri cittadini.

mi permetta di associarmi al dolore per tutte le vittime recenti e passate, perché realmente sentiamo che questa è una battaglia di civiltà. Impedire non solo le vittime, i morti, ma anche gli infortuni sul lavoro non credo sia un problema di una sola parte politica in quest'Aula. Ritengo che il lavoro, se viene fatto bene, troverà una larghissima condivisione da parte di tutte le forze politiche qui presenti. Tra le cose che lei ha annunciato e che farà, incontrando i vari rappresentanti del mondo del lavoro, così come del mondo dell'impresa, dell'università e delle varie organizzazioni che sono presenti nel territorio,

lavoro e una Commissione industria all'interno del Senato ed esistono anche delle professionalità (esclusa la mia) che potrebbero darle tanti buoni consigli nel suo lavoro. Per cui esiste al di fuori un mondo,

nel 2017. Chi muore si dà pace, si dice; ma avete pensato a chi rimane?

1.142 infortuni al giorno, che per fortuna non sono drammatici come quelli mortali. Sono numeri che portano ai circa 417.000 infortuni riconosciuti nel 2017 e ai circa 640.000 denunciati; probabilmente, nella differenza tra denunciati e riconosciuti potrebbe esserci forse anche qualcosa in nero, che si perde nelle statistiche. Quello che ancora è da tener presente sono i numeri: 90 milioni di giornate di lavoro perse, 90 milioni di giornate di lavoro perse, che colpiscono sicuramente la persona che non va a lavorare, ma colpiscono anche le nostre imprese. Pertanto, salvaguardando i lavoratori che hanno un infortunio, noi contribuiamo indirettamente anche a creare quella positività nell'impresa che è assolutamente un obiettivo che chiunque si interessi del suo Dicastero vorrebbe raggiungere. I pilastri su cui mi baserei per trovare una soluzione al problema della sicurezza nel mondo del lavoro sono l'informazione, la formazione, la prevenzione e la protezione.

Ministro, lei ha fatto, non solo oggi in quest'Aula, ma anche precedentemente (cosa assolutamente legittima in una campagna elettorale), una serie di narrazioni

Adesso bisogna vedere quali di queste narrazioni e di questi sogni riuscirà a realizzare. Da cittadino, devo dire che spero che siano tanti,

ma vorremmo esserne parte, ripeto, nel proseguire questa amabile e piacevole chiacchierata nelle nostre Commissioni parlamentari,

le risorse disponibili, i fondi per poter realizzare questi sogni. Signor Presidente, l'informativa che il ministro Di Maio ha illustrato rappresenta una volta di più l'incoscienza con cui negli ultimi anni una certa classe dirigente ha trattato il tema del lavoro. Le morti bianche, gli incidenti sul lavoro, il precariato che si fa invisibilità sociale, la disoccupazione, la competizione tra genitori e figli per strappare un contratto sono le caselle avvelenate di un neoliberismo che è diventato prima verbo e poi programma elettorale, laddove un tempo si parlava di socialismo. La parola «dignità», con cui il ministro e vice *premier* Di Maio impegna il Governo su materie inerenti al lavoro, diventa una parola carica di densità sociale, quindi carica di densità politica; una parola che si aggancia all'eco di quell'articolo 36 della Costituzione che parla proprio della dignità come limite invalicabile della retribuzione a favore del cittadino. Il vice *premier* Di Maio ha ricordato Salvatore Lombardo, morto in uno stabilimento Fincantieri. Già, Confindustria, che è sempre pronta a fare la maestrina, a indicare sempre le buone ricette, talvolta esponendosi anche a figuracce, come era successo con il suo centro studi allorquando aveva annunciato sciagure e catastrofi

su questo non ha niente da dire oppure tace, come tace tutte le volte in cui chiediamo trasparenza circa i nomi di quegli imprenditori che hanno preso i soldi dalle banche e non li hanno restituiti, forse per avventurarsi nelle privatizzazioni all'italiana? A proposito, colleghi, vi invito a pensare all'idea di ripristinare una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, in modo che facciamo anche luce sugli NPL. Il Ministro ha qui richiamato le aziende partecipate dallo Stato a essere un esempio di sicurezza sul lavoro. Esserlo significa controllare quella filiera di subappalti concessi a soggetti - spesso cooperative - che si trasformano in un vero e proprio campo di battaglia, dove ci si annienta per accaparrarsi un contratto o una paghetta purché sia. E così non va bene. Se permettete, provo un certo imbarazzo nel sentire che proprio dai banchi di sinistra arrivano le critiche sul reddito di cittadinanza, che spazza via il ricatto di quegli imprenditori che continuano a dire: o prendete questo contratto, o vi adeguate a questa paga, oppure fuori c'è la fila di disoccupati pronti a fare ciò che tu oggi non di stranieri illegali che sono molto più facili da minacciare. Il neoliberismo, accettato dal centrosinistra come primo attore o con il sostegno a Governi tecnici, ha fatto sì che il lavoro diventasse sinonimo di occupazione, ma lavoro e occupazione non sono assolutamente la stessa cosa: il lavoro che diventa lavoretto, come un po' è nel predicato della frontiera della *gig economy*, che, se non normata, se non normata, rischia di produrre un moderno feudalesimo. Bene quindi ha fatto il ministro Di Maio a imprimere un segno evidente e marcato sui *riders*, cioè sui fattorini che consegnano il cibo a domicilio. Non servono nuove leggi. Quelle che ci sono vanno rispettate per onorare la legge e il lavoro. Investendo in sicurezza si rispetta la legge e si onora il lavoro. Per questo, premiare anche fiscalmente chi investe in sicurezza serve molto di più che intervenire con altre La sicurezza è un fatto culturale e i cittadini lavoratori sono centrali.

stoppare l'inganno della pubblicità del gioco d'azzardo. *(Applausi La sicurezza parte dai diritti e dalla dignità. Andiamo avanti, signor Ministro, abbiamo ricominciato a camminare sulla strada giusta, la strada del lavoro vero.

colleghi senatori, membri del Governo, vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'ennesimo atto criminoso e intimidatorio perpetrato ai danni di un amministratore locale della Provincia di Foggia. Foggia. Venerdì scorso è stata incendiata, tra l'altro in pieno giorno, l'auto del sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo. Solo qualche giorno prima era stata incendiata l'auto di Domenico Rignanese, caposettore dello stesso Comune. Le indagini sono in corso, ma appare verosimile la matrice mafiosa dei due attentati che hanno avuto luogo in un Comune che era tornato al voto l'anno scorso, dopo essere stato sciolto per mafia.

Oggi voglio portare la mia solidarietà, quella del MoVimento 5 Stelle, e - sono sicuro di non sbagliare - anche quella dell'intera Assemblea, alle vittime di questi atti vigliacchi, dicendo loro che le istituzioni non li abbandoneranno e - anzi - faranno tutto quanto possibile e necessario. Questi due attentati erano stati preceduti, tra l'altro di qualche giorno, dall'omicidio - l'ennesimo - di un pregiudicato, questa volta a Vieste. Purtroppo, in Provincia di Foggia operano pericolosi e radicati sodalizi criminosi, la cui portata mafiosa è stata sottovalutata per troppi anni, i quali, proprio grazie a questa sottovalutazione, giorno dopo giorno, hanno rafforzato la propria presenza e il controllo militare sul territorio. In definitiva, negli ultimi anni si è costituita una nuova, forte e pericolosa identità criminosa, definita dall'*ex* procuratore antimafia la quarta mafia italiana. Questa quarta mafia si è, per così dire, specializzata in alcuni settori, divenendone *leader*, come ad esempio quello del traffico internazionale di hashish e marijuana e quello delle rapine alle banche e ai portavalori. Non cito le altre attività criminose, come il *racket* e le estorsioni. Questa quarta mafia ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue, più di 300 omicidi negli ultimi quarant'anni, l'80 per cento dei quali è rimasto impunito.

Assolutamente no. Io mi domando: a un partito che governa un Paese, che ha quattro presidenti di Regione e capoluoghi di Provincia, gli viene smontato un gazebo perché non c'era la casellina (per cui la colpa è del Comune), che poi noi siamo andati in Comune a barrare?

In risposta a una nostra mozione, il Comune ha detto che i parcheggiatori abusivi non danno fastidio. Stessa cosa, parlando di antifascismo e di razzismo, come mai nel Comune di Firenze dal 2005 ad oggi sono stati dati 8 milioni e 52.000 euro al campo rom di Poderaccio. Sapete benissimo cosa è successo poi: conflitto a fuoco di domenica pomeriggio e un ragazzo che stava andando a lavorare ci ha lasciato purtroppo la vita. Allora, mi chiedo, se razzismo è giustamente distinguere in base alla razza, perché quei soldi non vengono dati ad altre comunità?

Signor Presidente, intervengo ancora, come ha fatto ieri il collega Parrini, per sollecitare

In quell'atto ispettivo noi chiediamo al Ministro della giustizia di esprimere le proprie valutazioni su quanto riportato da alcuni organi di stampa e che è stato oggetto

da Esselunga e dal costruttore Parnasi, siano stati fatti ad associazioni legate alla Lega Nord, per evitare che un finanziamento diretto alla Lega, sui conti della Lega stessa, rientrasse nel provvedimento di sequestro di 48 milioni di euro disposto dal tribunale di Genova, per riportare ai cittadini ciò che è stato tolto loro per attività estranee alla finalità per cui quei soldi erano stati stanziati. Noi insistiamo per capire se è vero che, prosciugati i conti della Lega, per evitare il sequestro, vi siano stati fondi significativi, come risulterebbe da quelle inchieste, dirottati su altri canali per essere comunque utilizzati. Insistiamo perché è interessante - credo - per l'opinione pubblica, per questa Camera e per il Parlamento sapere cosa pensa il Ministro della giustizia. Credo sia importante capire le valutazioni, data la rilevanza del problema. Sarebbe, infatti, grave se si scoprisse che uno dei partiti di Governo si è reso protagonista di un raggiro come quello che, secondo «L'Espresso», sarebbe stato perpetrato ai danni dei cittadini.